finestra") ***Nota di aggiornamento al Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2007-2011***

Colleghi, la seduta è iniziata. ALBONETTI *(RC-SE)*. Signor Presidente, colleghi senatori, colleghe senatrici, la Nota di aggiornamento del DPEF è stata correttamente presentata, così come richiesto dalla risoluzione parlamentare di accompagnamento al DPEF stesso, discussa e approvata nel luglio scorso. La Nota, pur nella sua sinteticità, è da apprezzare per l'indicazione più equilibrata rispetto al DPEF dell'obiettivo del Governo: perseguire simultaneamente sviluppo, equità sociale e risanamento, il nocciolo del programma dell'Unione in materia di politica economica. Ciò detto, il nostro Gruppo mantiene, così come già affermato dal collega Tecce, un classico atteggiamento di "critica costruttiva" sulla strategia macroeconomica fin qui delineata dall'Esecutivo. Prima di motivare più analiticamente il voto del Gruppo RC-SE*,* che preannuncio favorevole, ci sia consentita una digressione sulla strategia comunicativa che ha caratterizzato la presentazione e la discussione della finanziaria. A pochi giorni dal suo varo, i sindacati, riferendosi a presunte pesantissime ipotesi di tagli nel comparto della scuola, parlavano di «macelleria sociale». All'indomani della sua approvazione da parte del Consiglio dei ministri, i pochi quotidiani in edicola titolavano: «Ecco la finanziaria di Carlo Marx». I più benevoli parlavano di «manovra scritta sotto dettatura» di Rifondazione. Nei giorni successivi, tutta la stampa di riferimento nazionale si interrogava, denunciava, analizzava la sconfitta del riformismo di fronte ad una trionfante sinistra radicale (ultimo, in ordine di tempo, Giannini, su «la Repubblica» di ieri). Siamo abituati ormai da troppe stagioni all'uso a mo' di megafono di editoriali e corsivi, ma oggi, in questa lettura forzata della complessità della finanziaria, riconosciamo qualcosa di più, e precisamente il tentativo di descrivere la finanziaria per quello che non è, e per riscriverla, eventualmente, per quello che si vorrebbe fosse. Molti ambiscono al ruolo di «dettatori», a partire da Confindustria. Ma quando, nei tempi recenti, le imprese hanno ottenuto tanto da un Governo come oggi, con la riduzione del cuneo fiscale? E perché il TFR, che è dei lavoratori e non delle imprese, dovrebbe essere a disposizione degli investimenti privati piuttosto che degli investimenti dello Stato? E dove è finito il rischio di impresa quando, di fronte alla massima disponibilità del sistema creditizio, come di recente affermato anche a Capri, si insiste nel voler utilizzare risorse diverse da quelle dell'autofinanziamento o, appunto, dal ricorso al credito? [**Presidenza del vice per l'economia, Edmund Phelps, su «Il Sole 24 ORE», qualche giorno fa, indicava proprio nella necessità di ricorrere al capitale di rischio una delle possibilità del sistema Italia. E, a proposito di "finanziaria marxista", come la mettiamo con l'aumento delle spese militari che noi chiediamo di ridurre o con i 1.000 milioni di euro previsti per le missioni? Si confrontino, da questo punto di vista, le proposte delle associazioni che hanno promosso la campagna «Sbilanciamoci», per verificare la distanza tra la nostra idea di finanziaria alternativa e quella proposta, che invece è, più propriamente, un tentativo di correzione delle distorsioni introdotte dal Governo precedente e delle profonde ingiustizie causate dalla politica economica di Berlusconi e Tremonti. Se poi ancora qualcuno avesse dei dubbi, si studi bene il rendiconto finanziario dell'anno 2005, che fotografa la difficile situazione dei conti dello Stato. Condividiamo l'impianto della finanziaria e, come ha detto bene il collega Tecce, l'aspirazione a coniugare risanamento, sviluppo ed equità, ma non rinunciamo, nel rispetto dei saldi ulteriormente definiti l'altro ieri dal ministro Padoa-Schioppa, a far sì che il Governo e la sua maggioranza recuperino a pieno il consenso sociale del Paese, migliore stella polare per la nostra navigazione che non i parametri finanziari e monetaristi della Comunità europea. Così oggi sottolineiamo con piacere il raggiunto accordo tra Governo ed enti locali, che destina quasi un miliardo di euro in più di risorse agli enti locali, ma chiediamo che queste risorse non siano sottratte ai lavoratori e alla spesa sociale; ci sono tutte le condizioni per farlo, come la Nota aggiuntiva suggerisce. La Nota, in effetti, indica una crescita economica italiana più sostenuta del previsto, probabilmente sottostimata se si è assestata all'1,2 per cento nel primo semestre 2006 ed è infine stimata solo allo 0,4 per cento nel secondo semestre. Indica altresì maggiori entrate fiscali: 6 miliardi di euro, di cui 5 strutturali; forse anche queste entrate sono state sottostimate. Questi dati ci confortano e, come già detto, confermano che l'idea da noi avanzata di una manovra più leggera e meno congiunturalmente legata alla riduzione del rapporto tra PIL e debito pubblico era praticabile e non irrealistica. All'opposto delle entrate, gli effetti negativi dovuti al calcolo dei rimborsi dopo la sentenza europea sulla detraibilità dell'IVA sono stati misurati nei loro valori massimali: 3.700 milioni di euro di minor gettito per il 2006 e maggiori oneri per 13.400 milioni di euro di rimborsi. Questo dato annulla la possibilità di ridurre l'entità della manovra, che rimane immutata, nonostante, come detto, l'andamento molto positivo delle entrate. Facciamo nostra la richiesta del senatore Morando al Governo affinché riferisca rispetto alla responsabilità politica del mancato riconoscimento da parte dell'Unione Europea del grave danno che la sentenza avrebbe causato alle finanze italiane. La nostra fiducia nella ripresa - che l'azione del Governo può aiutare e orientare non solo verso il recupero di competitività, ma anche verso il raggiungimento di più vere condizioni di equità anche, perché no, attraverso la rimodulazione delle aliquote IRPEF - ci permette di traguardare il raggiungimento pieno degli obiettivi complessivi del programma dell'Unione sull'intera legislatura. Il nostro voto favorevole alla Nota di aggiornamento è un viatico per far sì che continui il confronto sulla finanziaria, nel Parlamento e nel Paese, evitando promiscui per quanto volenterosi tavoli, affinché la finanziaria corrisponda nel modo migliore alle grandi e molteplici attese del Paese, a partire dal mondo del lavoro.

truffaldino. Prendo atto dello sforzo enorme e generoso con il quale ieri il presidente Morando ha cercato di giustificare ciò che il Governo ha scritto in questa Nota, ciò che il Governo ha scritto in questa Nota, che serve, come ho detto ieri, a nascondere all'opposizione, ma anche alla maggioranza, la realtà dei conti pubblici, in funzione di un'operazione politica che dovrà essere fatta nella prossima legge finanziaria. Ribadisco che una posta di stato patrimoniale non può essere messa in conto economico. Chiunque lo facesse compirebbe in questo Paese un falso in bilancio.

ripeto, cari colleghi, 18 miliardi di euro, emersi a seguito della sentenza della Corte dell'Aja sulla deducibilità dell'IVA - ad aumento del *deficit* pubblico del 2006. Non ad aumento del debito, quindi, essendo un debito pregresso, cioè nello stato patrimoniale, ma ad aumento del*deficit*, cioè nel conto economico.

serve a giustificare in un certo senso l'entità della manovra della legge finanziaria, ponendo a confronto la situazione 2005-2006 con la situazione 1992-1993. Cari colleghi, lungi da me sottovalutare le difficoltà della finanza pubblica italiana, avendo avuto modo, da trent'anni, di segnalare la china pericolosa con la quale i Governi dell'epoca

metà dell'attuale debito pubblico italiano si è formato in quegli anni: gli anni, ricordo, della solidarietà nazionale. fu nascosto agli occhi degli italiani, perché in quegli anni tassi di inflazione del 23-24 per cento nascondevano

Stato. I tassi di interesse, infatti, apparentemente elevati erano enormemente inferiori al tasso di inflazione. Fu un uomo di grande intelletto, di grande trasparenza, di grande coraggio politico, un cattolico, che si permise di richiamare l'allora massima potestà dello Stato del Vaticano a rispettare gli impegni finanziari. Fu una persona che è stata seduta su questi banchi per molto tempo, Nino Andreatta, che nel 1981, con il divorzio tra Tesoro e Banca d'Italia, fece scoprire l'inghippo. Dal punto di vista contabile, dunque, è solo dal 1981-1982 che il debito pubblico comincia a crescere in modo violento. In realtà - ripeto - metà di quel debito ha le sue radici nel periodo 1975-1980.

pur apprezzando la posizione anche di esimi ex colleghi economisti, come il professor Graziani e il professor Acocella, che hanno firmato un documento per la stabilizzazione.

gli interessi sul debito pubblico erano superiori al 12 per cento di PIL. Quindi, quell'1,8 per cento di avanzo primario del 1992 era a fronte

questi dati per una precisazione della storia. Ma perché il Governo insiste nel denunciare la gravità, la tragedia dei conti pubblici? Perché, in realtà, deve nascondere l'operazione che attuerà dentro la finanziaria, che a sua volta nasconde l'operazione vera che sta al di fuori e sopra la finanziaria. L'operazione presente nella finanziaria, che trova in questa Nota un timido senso di giustificazione con truffe contabili, è, quella sì, da un lato, di sanare il *deficit* pubblico, ma solo per 15 miliardi di euro. Gli altri 20 miliardi

- che in cinque anni la spesa pubblica corrente non è stata sufficientemente controllata dal precedente Governo. In cinque anni, però, essa è aumentata di due punti di PIL,

in quei 20 miliardi di euro; c'è solo un accentramento delle risorse nei singoli Ministeri; un aumento di 28 miliardi su 34 di entrate pubbliche. Al mio Paese queste si chiamano tasse. Tutto questo serve per tenere buona la sinistra estrema,

a intaccare le cronache di questi giorni: dagli accordi sulle fusioni bancarie ai tentativi di spostare fintamente la Telecom nello Stato. In realtà, attraverso la Cassa depositi e prestiti, la Telecom finiva nelle mani di chi avrebbe

che Garibaldi a Teano non diceva «Obbedisco» a quel piccoletto a cavallo che veniva dalla Savoia, ma a qualcun altro.

È ora di finirla con l'epoca del Britannia, e siccome casualmente c'ero, vi posso raccontare Signor Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, colleghi, sono bastati pochi mesi degli apprendisti stregoni per creare il caos nell'economia italiana. Avete iniziato voi a cambiare il rapporto con i contribuenti; il Grande fratello del decreto Visco-Bersani ha radicalmente cambiato il clima di fiducia fiscale che si era prima instaurato. Avete proseguito con la distruzione della fiducia dei mercati, iniziando con il crollo del mercato immobiliare (in una sola settimana fu bruciato un miliardo e 400 milioni); gli effetti sulla Borsa dell'operazione Telecom sono ancora visibili; recentemente il decreto collegato alla finanziaria ha cambiato il meccanismo di tariffazione dei pedaggi autostradali facendo crollare, anche qui, le prospettive di crescita delle società autostradali; avete previsto, in un decreto sugli affitti, che gli immobili cartolarizzati non possano essere rilasciati, in questo modo facendo crollare, ancora una volta, la fiducia nei mercati internazionali. In sostanza, grazie alla vostra azione di pochi mesi, è caduta la credibilità del sistema Paese nei mercati internazionali. *(Applausi accontentati di far cadere la credibilità all'esterno, l'avete fatto anche all'interno: preannunciando con mesi di anticipo la variazione della tassazione sulle rendite finanziarie, avete fatto scappare verso l'estero il risparmio italiano; con lo scippo di 5 o 6 miliardi del TFR non farete partire il risparmio previdenziale e la Borsa in Italia. Andate distruggendo ciò che di buono era già presente nel nostro Paese, ma questo non vi bastava, perché avete voluto proseguire con la legge finanziaria. La legge finanziaria sarà forse la causa di un peggioramento della ragione di *rating* del nostro Paese, cari apprendisti stregoni, dopo aver evocato la magia di un manovra forte, di una manovra fortissima da 35 miliardi, non siete stati in grado di rendervi conto che non era più necessaria una manovra di quell'entità; siete dovuti andare avanti perché questi erano gli impegni con l'Europa e adesso vi trovate nella difficoltà di realizzare una manovra irrealizzabile. Voi dite che i vostri predecessori avevano rovinato il bilancio, ma nella Nota aggiuntiva al Documento di programmazione oggi in esame riconoscete che i risultati del 2006 sono, a consuntivo, migliori rispetto a quelli che erano stati previsti nella finanziaria del precedente Governo. Volete che Bruxelles vi imponga una manovra fortissima, ma non avete le capacità di realizzarla; mi domando, signor Presidente, dove sono le riforme strutturali, dov'è la riduzione della spesa pubblica che avevate FI e del senatore Baldassarri).* Vi vantate di avere il consenso della sinistra e della sinistra estrema - gli *slogan*, d'altronde, sono della sinistra estrema - ma non avete avuto il coraggio di chiedere in cambio riforme strutturali, soprattutto nel settore delle pensioni e del pubblico impiego. Voi cavalcate la rivoluzione per via fiscale, ma non siete in grado di ottenere null'altro. Dite che la vostra manovra è improntata allo sviluppo, ma si tratta di una manovra che non porterà ad altro che ad una recessione ulteriore del sistema economico. Dite che poche sono le tasse previste in questa manovra, solo 5 miliardi, ma, come dimostrano gli economisti di sinistra, le tasse, tra vecchie e nuove - si parla di 67 nuovi balzelli aggiuntivi - sono circa l'80 per cento della manovra, almeno 25 miliardi di euro, miliardi di vecchie lire. Dite che siete a favore del mercato e del cittadino - questa sarebbe la vostra filosofia Bersani ma, in realtà, nei più di 100 articoli aggiunti l'ultima notte, forse dopo l'approvazione da parte del Consiglio dei ministri del testo della finanziaria, vi occupate esclusivamente di fare elargizioni a vostri settori di collateralismo politico e create dei costi che tolgono risorse ai cittadini, facendo pagare loro più tasse. Dite che farete piangere i ricchi e tassate i poveri, se è vero, come ha dimostrato un quotidiano economico assolutamente non vicino alla nostra parte politica, che la tassazione, tra variazione dell'aliquota IRPEF e addizionali comunali e regionali, che voi regalate a larghe mani agli enti decentrati, inizia a mordere già per un lavoratore con coniuge a carico e due figli a partire da un reddito di 20.000 euro lordi annui, cioè poco più di 1.000 euro netti al mese. Se questi sono i ricchi, complimenti per la visione della società che voi avete. Dite che volete pacificare il Paese e intanto non fate altro che fomentare l'invidia sociale come metodo di Governo. Ma vi è mai passato per la mente, signor Presidente, che la produzione sia essenziale prima della redistribuzione? Che senza produzione non esiste redistribuzione e che, come dice il Ministro degli affari esteri, forse è meglio far sorridere i poveri che far piangere i ricchi? Dite che volete diminuire il costo del lavoro e che quindi volete intervenire sul cuneo fiscale, ma intanto aumentate i contributi sociali in misura elevatissima per i lavoratori autonomi e li aumentate anche per gli stessi lavoratori dipendenti. Ma quale è la coerenza che vi guida in questa azione? Dite che volete spalmare il cuneo fiscale anche per la parte dei lavoratori; il 40 per cento deve essere restituito ai lavoratori, ma lo fate - basta leggere la Relazione previsionale e programmatica - non restituendo a ciascuno il suo, ma con la modifica della curva dell'IRPEF. In sostanza, togliete ai lavoratori di stipendio medio e medio-alto la loro parte di cuneo fiscale, dandola ai ceti più deboli, ma anche a chi non lavora, a chi non ha mai lavorato, a chi ancora non lavora

Dite che volete rendere funzionale la pubblica amministrazione e intanto cacciate tutti i dirigenti solo per fare prevalere una logica di*spoils system*, che vuole semplicemente consentirvi di impadronirvi di tutte le leve del potere. È questo il buon funzionamento della pubblica amministrazione? Dite che vi sentite più vicini all'Europa, che questo finalmente è un Governo europeista e intanto stracciate la realizzazione delle grandi opere infrastrutturali cofinanziate dai fondi pubblici. Basti pensare all'alta velocità o al ponte di Messina; questo modo permettete che non solo non si realizzino le opere pubbliche in Italia, ma che i finanziamenti che sarebbero stati destinati a noi saranno distratti a favore di altri Paesi europei. I cittadini italiani pagano e gli altri viaggiano meglio. Dite che non volevate ripristinare la tassa di successione e donazione e invece, nel decreto fiscale, l'avete ripristinata semplicemente chiamandola

che siete favorevoli alla tutela del risparmio e intanto, come dimostra la delega fiscale collegata alla finanziaria, avete deciso di aumentare la tassazione sui BOT, sulle obbligazioni, sugli altri titoli finanziari e anche, come è espressamente sancito all'articolo 1, sul circolante, quindi su tutti i titoli già emessi. Voi tassate quindi di più il risparmio degli italiani e, con l'aumento delle rendite catastali, anche le loro case. Li state gradualmente espropriando nel loro patrimonio. Dite che la manovra finanziaria è perfetta, il ministro Padoa-Schioppa ha detto che bisogna prendere o lasciare, e intanto non si contano gli errori e le marce indietro che state facendo.

bonapartista di un vero e proprio regime. Signor Presidente, la luna di miele tra il Paese e il Governo è subito finita. Anche molti dei vostri elettori si sono già pentiti; siete riusciti in un vero miracolo politico, ma è un miracolo che si sta tramutando in una vera e propria tragedia per il Paese. Per questo annuncio il voto favorevole di Forza Italia alla risoluzione n. 1.

con la Nota di aggiornamento al DPEF affrontiamo dei temi cruciali per il Paese: il rilancio dello sviluppo economico e il riequilibrio delle condizioni di vita che per molti italiani, troppi, sono peggiorate nel corso dell'ultimo quinquennio. Colleghi, il tema è talmente pressante nella scala delle priorità che sarà necessario trovare delle convergenze, tanto nell'analisi, quanto, possibilmente, nelle soluzioni, dal momento che i problemi di cui stiamo trattando sono seri e meritano di essere affrontati non già con un'arma contundente per difendere le proprie posizioni, ma nell'ottica di una preziosa occasione per un confronto politico. Nel corso del dibattito,

che l'opposizione può dormire sonni tranquilli: noi non abrogheremo questo reato, né lo modificheremo ad uso e consumo nostro. Argomentare una tesi con i numeri è cosa differente, è cosa più impegnativa, significa farlo con la logica della matematica e non con l'arte oratoria. I numeri non sono né pessimisti, né ottimisti, né di destra, né di sinistra, sono numeri che ci aiutano a capire la realtà e ad intervenire per correggerla. È proprio questa ragione dei numeri che emerge in modo evidente dalla Nota aggiornamento al DPEF ed è sufficiente analizzarla con onestà intellettuale per cogliervi una favorevole evoluzione dei parametri economici. Ne indico quattro, senatore Vegas.

a rivedere lievemente al rialzo la stima della crescita per il 2006 (all'1,6 per cento, rispetto all'1,5 indicato nel DPEF). Il terzo è l'aumento delle entrate tributarie erariali, valutabili per il 2006 in un gettito maggiore di circa 6 miliardi rispetto a quanto previsto; circostanza, questa, che permetterà di contenere l'entità della manovra necessaria. Quarto, il debito in rapporto al PIL, senatore Baldassarri, che, previsto in graduale riduzione fino ad arrivare all'obiettivo del 97,8 per cento renderà più sostenibile il risanamento indicato dal Consiglio ECOFIN del luglio 2005 e, cioè, la riduzione di quell'indebitamento netto di 1,6 punti percentuali nel biennio 2006-2007 e l'aumento di quell'avanzo primario cento entro il 2011. Questi sono numeri, colleghi, non chiacchiere, non opinioni. Spesso i nostri dibattiti, signor Presidente, sono affetti da un vizio tipico della politica: non si parla del documento in esame, ma di altro. Ma è questa ragione dei numeri

La vera novità della Nota in esame è il terzo dei punti che ho appena indicato, vale a dire il maggior gettito erariale (circa 6 miliardi per il 2006), depurato dagli effetti della congiuntura economica. Ilfattore positivo rispetto al passato risiede proprio nella circostanza che tale gettito è ascrivibile non solo all'attuazione delle misure previste dalla finanziaria 2006, ma è dovuto soprattutto ad un nuovo atteggiamento dei contribuenti i quali, verosimilmente, hanno ritrovato quella convergenza di interessi - venuta meno, negli ultimi anni, a causa dei ripetuti condoni fiscali introdotti dal centro-destra - mediante la quale hanno preso atto del fatto che il nuovo Governo e la maggioranza che lo sostiene operano nell'esclusivo interesse generale del Paese e non di una sua parte limitata. Senatore Vegas, da apprendisti stregoni è stato esattamente il tentativo della destra di accreditare le ripetute operazioni di finanza creativa per interventi strutturali: le numerose *una tantum*, l'alienazione degli immobili di Stato, i condoni edilizi, i concordati e le numerose operazioni di ingegneria contabile hanno prodotto piccole boccate di ossigeno nelle esangui casse dello Stato, ma ancora oggi ne paghiamo il prezzo in termini di maggior debito pubblico e, quel che è peggio, senatore Vegas, di sospetto con il quale non solo Bruxelles, ma anche le agenzie di *rating* osservano e giudicano il nostro operato. Ora, invece, i recenti segnali provenienti dal Fondo monetario internazionale e dal commissario Almunia sono senz'altro più incoraggianti. Detto ciò, non mancano elementi problematici, onorevoli senatori. Il primo è connesso alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee in materia di detraibilità dell'IVA sulle autovetture di servizio. Gli oneri derivanti da tale sentenza saranno particolarmente gravosi per i motivi ormai noti. Nel 2006 avremo un minor gettito di circa 3.700 milioni e 13.400 milioni di maggiori oneri per il pagamento degli arretrati relativi al 2003-2005. Non nascondiamo l'impatto di tali impegni sopravvenuti che, in certa misura, finiscono per ridimensionare il dato positivo del cresciuto gettito erariale. Ma come possiamo non ricordare che le misure contenute in questa sentenza erano state sollecitate dalla stessa Commissione europea sin dal 2005 e che il precedente Governo le ha deliberatamente eluse, rinviandone i pesanti oneri a partire da questo esercizio finanziario?

alcun controllo durante la scorsa legislatura. È su tali elementi che rimane altissima la vigilanza delle autorità europee, dei mercati internazionali e della nostra maggioranza. Il nostro Paese ha alle spalle un intero lustro caratterizzato da una crescita economica inferiore all'1 quasi come Grecia e Portogallo, la più bassa. Degli ultimi tre anni due sono stati caratterizzati da una crescita zero del prodotto interno lordo. C'eravate voi al Governo, non noi. Il rapporto *deficit**-*prodotto interno lordo è oggi al 4,6 per cento e deve rientrare al 2,8 per cento. L'avanzo primario è sostanzialmente scomparso, mentre nel 2005 risultava del 5,5 per cento. Negli ultimi tre anni il debito pubblico si è nuovamente impennato dopo una fase di progressiva, sia pur lenta, ma costante diminuzione cui l'avevano condotto i Governi di centro-sinistra: con il risultato che ora più della metà di ciò che entra nelle casse dello Stato è già ipotecato per coprire i debiti pregressi. Questi sono numeri, colleghi senatori, di cui il Governo Prodi è stato costretto a prendere atto: numeri difficili da smentire. A voi, colleghi della destra, resta la facoltà di avvalervi del diritto di continuare a fingere di non vedere e di non voler capire, se è così che pensate di fare l'interesse del Paese. II percorso inaugurato lo scorso luglio, con il DPEF è incentrato su tre obiettivi: crescita economica, risanamento, equità. Senza questi obiettivi, è l'intero ciclo di sviluppo del Paese che non potrà ripartire. È per questo, signori colleghi, signor Presidente, che l'Ulivo esprime un fermo e convinto sostegno al Documento oggi in esame perché anche noi, come insegna Kant, dobbiamo avere l'ambizione di cambiare le cose. Non possiamo e non vogliamo permetterci il lusso d trasmettere la paura del nuovo. Questa maggioranza è determinata a scrivere una bella pagina della nostra storia. E ci riuscirà, perché ha piena di fiducia nelle energie del nostro Paese!

ho avuto l'onore di conoscerlo. Rammento una lettera che mi inviò anni fa e ciò mi impone di ricordarlo, sia pure rapidamente. Matteucci è stato

L'anno scorso è uscito un suo saggio sul liberalismo che è davvero un testo da leggere e conservare. Era un liberale schietto; ha avuto una vita, soprattutto in età giovanile, piuttosto difficile. Il padre, come è ricordato oggi su «la Repubblica», fu vittima di una vendetta di classe nel 1945. Era un liberale davvero schietto che ci lascia esempi

A me interessava soltanto lasciare questo ricordo agli atti parlamentari. Informo che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha comunicato che nella seduta dell'11 ottobre 2006 ha verificato non essere contestabili le seguenti elezioni e, concorrendo negli eletti le qualità richieste dalla legge, le ha dichiarate valide: per la Regione Piemonte: Alfonzi, Benvenuto, Calderoli, Davico, Eufemi, Fluttero, Ghigo, Malan, Martinat, Menardi, Morgando, Negri, Piccioni, Rame, Tibaldi, Scarabosio, Stanca, Turco, Vegas, Vernetti e Zanoletti.

in qualità di Presidente della Commissione finanze e tesoro, riferisco sui lavori della stessa in ordine al disegno di legge n. La Commissione finanze e tesoro ha esaminato in tre sedute il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 258 del 2006, svolgendo un approfondito dibattito sui contenuti del provvedimento, anche in relazione alle proposte di modifica predisposte dalla relatrice, senatrice Thaler. Il valore tecnico dell'analisi compiuta,

Prego i colleghi dalla parte sinistra e anche da destra di lasciare l'Aula se non intendono ascoltare e di proseguire fuori le loro conversazioni. Non è possibile continuare a lavorare in questo modo.

stante la parità numerica dei componenti dalla Commissione finanze e tesoro, tutti gli emendamenti presentati sono stati respinti e non è stato conferito il mandato alla relatrice di riferire favorevolmente in Assemblea. Auspico, signor Presidente, che l'Aula possa consentire di riprendere il filo della discussione, anche apportando alcune modifiche migliorative, in accordo con la relatrice e il rappresentante del Governo.

Signor Presidente, come già evidenziato nella relazione all'Aula del Presidente della 6a Commissione, senatore Giorgio Benvenuto, oggetto della conversione in legge del decreto-legge 15 settembre 2006, n. 258, è l'attuazione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 14 settembre 2006 nella causa C‑228/05.

della direttiva 77/388/CEE. La Corte di giustizia prevede infatti che tutti gli Stati membri siano tenuti a conformarsi alla VI direttiva. Infatti, nel caso in cui un'esclusione dal regime delle detrazioni non sia stata stabilita in conformità all'articolo 17, n. 7, le autorità tributarie nazionali non possono opporre a un soggetto passivo una disposizione che deroga al principio del dritto alla detrazione dell'IVA, enunciato, appunto, dall'articolo 17, n. 1, della stessa direttiva. La decisione della Corte di giustizia delle Comunità europee ha dichiarato pertanto l'incompatibilità con i princìpi comunitari relativi alla detrazione dell'IVA

l'IVA sostenuta sulla spesa in questione è detraibile quando ne sussistano i requisiti dell'inerenza della spesa a operazioni imponibili relative al precipuo esercizio dell'attività d'impresa.

servizi importati o acquistati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione. Va peraltro fatto rilevare all'Assemblea che la Corte di giustizia ha contestato allo Stato italiano la violazione dell'obbligo procedurale, previsto dalla direttiva CEE in materia di imposta sul valore aggiunto, concernente la consultazione dell'apposito Comitato nei casi in nei casi in cui si intenda adottare una misura nazionale che deroghi al regime generale delle detrazioni dell'IVA. Ancora, sempre con riferimento alla predetta sentenza, corre l'obbligo ricordare che la norma censurata in sede comunitaria è stata introdotta nella legislazione italiana nel 1979 come misura permanente e solo dal 1980 è stato fissato un limite temporale di efficacia, sistematicamente prorogato.

a mio parere, in violazione degli obblighi comunitari, non abbia concordato la misura e le condizioni della proroga del regime di indetraibilità. in esame il Governo si è quindi proposto - a mio avviso - di dare attuazione alla più volte citata sentenza, mostrando, nello stesso dibatto che si è svolto in Commissione, particolare attenzione alle sollecitazioni, osservazioni e proposte formulate dalla stessa opposizione. Su questo versante si sono posizionate le stesse forze di maggioranza, proponendo, con riferimento al testo originario del decreto-legge, sicura attenzione verso le esigenze dei contribuenti e la necessità di non assegnare carattere decadenziale ai termini per la presentazione della eventuale domanda di rimborso. In questa logica si è mosso e si muove l'emendamento presentato in Commissione dalla senatrice Thaler e ora all'attenzione

per un termine di equilibrio da fissare fra le esigenze dei contribuenti e l'attenzione ed il pieno rispetto delle istanze dell'Unione Europea. Ritengo, quindi, che la stessa discussione che stiamo svolgendo possa proporsi l'obiettivo di addivenire ad una valutazione concorde, tenuto conto in particolare del fatto che l'emendamento proposto dalla senatrice Thaler, peraltro condiviso dallo stesso rappresentante del Governo in Commissione, risulta migliorativo del testo del decreto, laddove prevede la facoltà per il contribuente di scegliere tra la richiesta di un rimborso forfetario, secondo un regolamento attuativo che tenga conto dell'utilizzo della detraibilità dell'IVA differenziata per settori di attività, attività, in accordo con l'Unione Europea, e la possibilità di un rimborso integrale di quanto eventualmente indebitamente versato. A ciò si accompagna il fatto che il termine per la presentazione dell'istanza, come detto, non ha più natura decadenziale e viene spostato al 15 aprile 2007, dando così modo ai contribuenti di valutare quale sistema scegliere. Vi sono quindi - a mio avviso - le condizioni per addivenire ad un soluzione condivisa, tenendo conto, inoltre, del fatto che il decreto-legge correlato alla manovra finanziaria per il 2007 contempla una disposizione che modifica il regime ai fini IRPEF e IRAP dell'IVA detraibile, a partire dall'anno di imposta 2007, mentre per il pregresso intervengono le norme che l'Aula è chiamata a discutere e ad approvare. *(Applausi

decreto-legge in esame, in quanto le disposizioni da esso recate, contrariamente alle finalità enunciate dal Governo, di dare seguito alla sentenza della Corte di giustizia europea, definiscono modalità e condizioni a dir poco subdole ed impossibili per ottenere il rimborso dell'IVA indebitamente pagata ed avranno un effetto assolutamente penalizzante per i contribuenti italiani interessati dalla norma. Al di là dell'incertezza circa la quantificazione del rimborso che i contribuenti dovranno richiedere, è evidente che l'esclusione dell'utilizzo della compensazione e della detrazione spettante confligge con la disciplina comunitaria. Pertanto, questo decreto dovrà essere ricordato, nel caso in cui lo approverete, e considerato come un raggiro del Governo ai danni delle categorie interessate. Bene ha detto il collega Pegorer, effettuando una disamina sotto l'aspetto della normativa comunitaria, che questo provvedimento è assolutamente in contrasto, come rimborso, con quanto stabilito con sentenza dell'11 maggio 2006 dalla Corte di giustizia. Infatti, proprio in relazione alla concessione governativa e ai rimborsi per l'iscrizione nel Registro delle imprese la Corte di giustizia condanna giustizia condanna tutte le restituzioni che subordinano il tributo dichiarato incompatibile con il diritto comunitario da una sentenza della Corte (incompatibilità dunque espressamente dichiarata) ad una norma di rimborso sfavorevole alle parti interessate.

affermando l'incompatibilità della disciplina IVA nazionale in materia di detrazione dell'IVA relativa alle auto aziendali con la VI direttiva in materia IVA. Quando nasce la storia? La direttiva risale niente meno che al al 1977 e, nella sua sostanza, la disciplina nazionale su questa materia è invece del 1980. La direttiva stessa consentiva di escludere dal regime di detrazione

L'Italia ha provato addirittura ad affermare che tale esclusione era motivata con cause di tipo congiunturale che risalgono al 1980, cioè da una congiuntura durata oltre un quarto di secolo. La cosa si fa più imbarazzante quando arriviamo a tempi a noi più vicini, perché, a fronte dell'accendersi della discussione intorno alla francamente evidente incompatibilità della disciplina nazionale con la disciplina comunitaria, il Governo italiano, nel 1990 prima e poi ancora nel 2000,

per cinque anni ha governato il centro-destra; l'Italia non ha mantenuto gli impegni e la decisione della Corte a quel punto si faceva probabilmente scontata. lunga storia di inadempienze e anche di leggerezza del Governo italiano nel suo complesso (ripeto, la storia parte dal 1980) nel confrontarsi con le regole del mercato comune. c'è una parte più imbarazzante sulla quale vorrei richiamare l'attenzione in questa Aula. La sentenza con la quale la Corte di giustizia ha affermato l'incompatibilità tra la disciplina nazionale sull'IVA e la VI direttiva

(diciamolo brutalmente) vale per il futuro e non per il passato, perché se si consentisse alla stessa, come di norma dovrebbe essere, di produrre effetti anche con riferimento al passato, lo Stato membro potrebbe ricavarne grande danno. La Corte, pur ribadendo questo principio,

"il Governo italiano non è riuscito a dimostrare l'affidabilità del calcolo in base al quale esso ha sostenuto dinanzi alla Corte che la presente sentenza rischierebbe, qualora i suoi effetti non fossero limitati nel tempo,

Corte afferma di non aver acconsentito alla richiesta di limitare gli effetti temporali perché il Governo italiano non ha prodotto informazioni affidabili, in grado di dimostrare la rilevanza di tali effetti.

nelle istituzioni), non presentando conti affidabili alla Corte, ha consentito che si producesse un danno per l'erario, e quindi per il contribuente italiano, di 27.000 miliardi Il danno può essere stato determinato da negligenza o incapacità nella difesa, o da negligenza o incapacità in capo a coloro che avrebbero dovuto fornire a chi rappresentava l'Italia davanti alla Corte gli elementi di fatto necessari.

approvare il decreto-legge, con il quale - ripeto - si dà attuazione alla sentenza e si garantiscono ai cittadini italiani diritti che essi hanno in virtù della sentenza medesima, necessario e doveroso da parte del Governo procedere ad una formale indagine amministrativa, per verificare in capo a chi collocare la responsabilità di quanto la Corte afferma solennemente nella sua sentenza. Non è immaginabile che i contribuenti italiani subiscano un danno di 27.000 miliardi di vecchie lire (un punto di PIL: per capirci, circa l'entità complessiva della manovra finanziaria netta, ovviamente quella rilevante, relativa alla correzione dei conti pubblici, che discuteremo in queste Aule nei prossimi mesi) e non si accertino le responsabilità eventuali, relative ad inadeguatezza, incompetenza, insufficienza e negligenza. Pertanto, nel ribadire il nostro sostegno al decreto all'attenzione del Senato, chiediamo e continueremo a chiedere al Governo di avviare una formale indagine amministrativa per accertare la responsabilità che ha prodotto questo danno.

colleghi senatori, stiamo discutendo di un decreto emanato in conseguenza ad una opportuna decisione della Corte di giustizia delle Comunità europee, che ha dichiarato l'incompatibilità delle norme italiane in merito alla indetraibilità dell'IVA per gli autoveicoli, per i servizi e per i mezzi di consumo relativi a questi strumenti. Al di là della incertezza circa la quantificazione del rimborso che i contribuenti potranno e dovranno richiedere, è evidente che il principio fondamentale che soggiace alla necessità di fornire compiuta risposta alla sentenza dell'Unione Europea, e quindi di vedere soddisfatte le esigenze dei contribuenti italiani, non è attuato. Non viene data esatta applicazione a questo principio fondamentale, in particolar modo, per quanto prevede questo decreto, con l'esclusione dell'utilizzo della compensazione e della detrazione spettante al contribuente. Tale impedimento confligge con la disciplina comunitaria. Noi potremmo anche, come abbiamo fatto in Commissione finanze, esaminare brevemente i due commi dell'articolo uno che compongono e sostanziano il decreto. Potremmo in questo caso informarci della fondatezza delle mie premesse, cioè del fatto che questo decreto poco e male dà risposta alle opportune e giuste aspettative del contribuente. Il comma uno è una somma di indeterminatezza e di approssimazione. Si pensi all'invio delle domande di rimborso in via telematica, le cui difficoltà sono già state evidenziate e discusse sin dall'esame del decreto Bersani-Visco: la data del 15 dicembre per la presentazione delle domande,

opportuna in linea di principio ma assai complessa nella contabilizzazione, della ponderazione dell'insieme dei benefici, la detrazione IVA, e costi, cioè la conseguente imponibilità ordinaria fiscale relativa ai minori ammortamenti. Questa stessa

preclude l'utilizzo delle generali procedure di detrazione e compensazione dell'IVA disciplinate dalla legge n. 633 del 1972 che costituisce questo tipo d'imposta. Per essere breve, e nonostante i ragguardevoli paletti introdotti in questo decreto, comunque l'erario dovrà restituire somme ragguardevoli al contribuente: poco fa era citato questo problema. problema. I dati di aggiornamento al DPEF, e questo aspetto è stato valutato anche in questa sede, mostrano che dovremo scontare un minor gettito di 3.700 milioni di euro per il 2006 e maggiori oneri, pari a 13.400 milioni di euro, per il pagamento degli arretrati per gli anni 2003, 2004 e 2005. e 2005. Sembra che tutto si concluda con un ostruzionismo da parte di un decreto, e quindi della maggioranza e del Governo, ai diritti dei contribuenti.

di attribuzione dei valori, ai fini della contabilità, della autovettura data in uso ai dipendenti. Si tratta di una serie di norme che va nella direzione di

«La presente relazione intende stimare l'effetto a regime sul gettito delle nuove disposizioni che ai fini delle imposte sul reddito decorrono dal 1° gennaio 2006. Nel primo paragrafo viene stimata la perdita di gettito a regime della detraibilità IVA conseguente alla Sentenza della Corte di Giustizia del 14 settembre 2006. Nel secondo paragrafo viene stimato l'effetto di compensazione a regime della nuova norma». Tutti i discorsi che facciamo sulle responsabilità politiche di chi non ha detto che la sentenza della Commissione di giustizia europea avrebbe avuto grandi rilievi ed incidenze sulla finanza pubblica italiana, sono discorsi solamente di merito, strumentali, sono stati fatti tanto dal presidente della Commissione bilancio, il collega Morando, ma anche oggi poco fa dal senatore D'Amico, perché nella sostanza si crea una risposta altrettanto costosa, naturalmente per le casse dei contribuenti, togliendo con la mano sinistra quello che si deve dare oggi con la mano destra. Chi parla di grave danno finanziario al bilancio pubblico italiano ha ragione: parliamo di cifre molto rilevanti (15 o 20 miliardi di euro) però, signori miei, queste sono somme che sono state evidentemente sottratte in maniera arbitraria dall'erario italiano ai contribuenti, cioè agli imprenditori, a quelli che sono il motore della nostra economia. allora, prima di chiedere al Governo di fare un'indagine sulle responsabilità della mancata ottimale difesa degli interessi pubblici italiani (italiani nel senso dell'erario, nel senso dello Stato), forse bisognerebbe pensare chi mai ha difeso gli interessi del contribuente; in questo caso vi è l'ulteriore dimostrazione che gli interessi del contribuente contribuente non sono mai difesi, perché, come ho dimostrato e spiegato, con un decreto si toglie quello che si dà con l'altro. Si svela allora quest'arcano: in barba alle disposizioni della Corte di giustizia europea c'è questa contromossa.

l'azione fiscale tributaria della pubblica amministrazione in senso estensivo, quando si tratta di sostenere il livello del prelievo, e restrittivo quando si tratta di garantire uniformità, chiarezza e certezza delle norme applicate. Non trovo altra giustificazione a questo comportamento.

ha presentato e ripresentato degli emendamenti in modo di cercare di avvicinare il testo del decreto ad una applicazione più concreta e certa, cosa che invece, come ho detto all'inizio, non avviene oggi. Ritengo comunque - ne discuteremo in sede di esame degli emendamenti - che neanche quell'emendamento dia le risposte di chiarezza e di certezza del diritto tributario che il contribuente penso abbia assolutamente

sentenza della Corte di giustizia europea, di cercare di ragionare su delle soluzioni comuni che vadano nella direzione di dare davvero queste risposte.

riferire in Aula, mentre alla Camera poi invece, con altri decreti, si fa quello che dicevo prima: un aggravio contributivo in modo da annullare il beneficio della detraibilità dell'IVA. Se queste sono le condizioni del dialogo e della discussione

voglio farlo in senso positivo e propositivo. Se è impossibile, per quanto riguarda voi e per quanto riguarda noi, aderire a qualche proposta che giunga dall'una o dall'altra parte, visti gli anni luce che ci separano su temi come quello oggetto del dibattito odierno, perché non vi confrontate con le categorie economiche interessate, quando assumete decisioni di particolare rilevanza, come quelle dei due decreti che ho delineato in questa sede? Allora, se all'interno di quest'Aula e della nostra Commissione non ci sono le condizioni politiche - penso di averlo ben ampiamente giustificato - ci sia almeno la dignità, per evitare di

presenti sul tappeto. Dovreste avere l'onestà di intenti di ragionare con loro delle date, delle scadenze e dei termini di rimborso, delle compensazioni, naturalmente dovrebbero essere frutto di una opportuna concertazione. Ma neanche questo è fatto, però dimenticavo - l'ho detto poco fa - che se questo è espresso come linea di principio, forse non è un diritto di cui godono i «sudditribuenti» italiani che sono quelli che devono solo pagare e non hanno grandi diritti ai tavoli di trattativa.

sotto questo profilo, sappia discutere e approvare emendamenti validi e proficui; mi auguro che ci renda conto che la filosofia

che viene presentato in Aula senza il mandato al relatore dimostra la debolezza di una maggioranza che non riesce neppure ad assolvere a questo compito. compito. Nonostante queste condizioni di difficoltà, la stessa maggioranza si è arroccata nella difesa di un decreto francamente indifendibile. Il senatore D'Amico ha poi introdotto un ulteriore elemento come il comportamento del Governo italiano nell'azione di difesa; certamente questa è una posizione non condivisibile, anche perché quelle stesse argomentazioni avrebbe potuto dirle, esplicitarle direttamente in Commissione, chiedendo al Ministro dell'economia e delle finanze o al vice ministro Visco di venire a riferire su questa questione o anche al Ministro per le politiche comunitarie. Avremmo avuto tutte le notizie e le informazioni necessarie. Questo non è stato fatto, evidentemente soltanto per introdurre un elemento di polemica che non ha ragione di esistere. Questo decreto è la prevedibile, onerosa conseguenza di atti normativi nazionali in materia di IVA adottati nel tempo, in totale contrasto con i princìpi comunitari. Alla chiara pronunzia della Corte di giustizia relativa alla detraibilità dell'IVA per acquisti di autoveicoli nella sussistenza dell'inerenza della spesa e della afferenza all'esercizio dell'attività di impresa, il Governo ha risposto con un decreto confuso, vago, opaco nelle modalità applicative, teso ad evitare ogni obbligo, così come ha fatto introducendo norme nel decreto-legge n. 262 che vanificano, appunto, la sentenza europea. europea. Non è questa la sede per individuare responsabilità risalenti nel tempo, ma che apparivano chiaramente in contrasto con inequivocabili princìpi comunitari, adottati proprio per evitare che un'imposta come l'IVA possa costituire un mezzo che alteri la parità degli operatori economici nell'Unione Europea. Europea. Il primo problema che abbiamo di fronte è quello della copertura del decreto. Nella relazione di accompagnamento viene detto esplicitamente che il provvedimento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Come può avvenire tutto questo, come si può dare esecuzione ad una sentenza senza i relativi oneri? Siamo invece in presenza di sentenze internazionali che vanno equiparate a sentenze interne onerose e, quindi, per l'obbligo di compensazione rispetto alla contabilità nazionale. Le previsioni, dunque, non sono corrette, poi, perché le disposizioni avrebbero dovuto essere abrogate. Conseguentemente, i soggetti di imposta IVA potranno portare in detrazione l'imposta pagata in via di rivalsa sugli acquisti delle autovetture.

oggettivo, che debba farsi ricorso alla prescrizione ordinaria. Questo invece non accade, perché il Sottosegretario si è arroccato nella possibilità di detrazione dal periodo di imposta 2003. Voglio aggiungere ancora che la giustizia europea non ha accolto le motivazioni italiane sul danno grave per l'erario, soprattutto perché non era una misura temporanea o congiunturale, ma di adattamento strutturale del sistema non giustificabile. C'è un'altra perla in questo decreto: viene introdotta una procedura speciale che preclude l'utilizzo delle generali procedure di detrazione e compensazione disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica n. 633, e rappresenta un altro grave limite alla detrazione riconosciuta dalla Corte di giustizia. Profili di incompatibilità comunitaria, dunque, presenta anche la modalità prevista per il rimborso perché il principio di equivalenza, il principio di conservazione degli effetti delle pronunce e il principio di effettività con modalità che ne rendano impossibile o eccessivamente gravoso l'esercizio del diritto vengono di fatto preclusi.

Questo decreto non è altro che nebbia che piomba sulle imprese, impedendo qualsiasi navigazione certa, e che pone problemi seri rispetto alla certezza dei bilanci delle imprese. Signor Presidente, dobbiamo dare atto, al presidente Manzella e alla Commissione Politiche dell'Unione Europea, di aver predisposto un parere che possa e debba essere tenuto in debita considerazione. Il Gruppo UDC, attraverso specifici emendamenti, ha operato in senso costruttivo, guardando prioritariamente a dare concreta esecutività alla pronuncia europea e a creare migliori condizioni per i contribuenti in termini di recupero delle somme non dovute all'erario. Per queste ragioni riteniamo si debba intervenire sul corpo del decreto-legge. Occorre necessariamente prevedere l'allungamento dei tempi di scadenza delle domande, troppo ravvicinati e inadeguati rispetto ai principi dello Statuto del contribuente tante volte richiamati e sempre disattesi e prevedere altresì le compensazioni fiscali, giacché la procedura speciale preclude l'utilizzo della generale procedura di detrazione e di compensazione, rappresentando un ulteriore grave limite. inoltre, la presentazione delle domande nelle diverse forme e, dunque, non soltanto in via telematica, rendendo valide anche quelle presentate nei termini e consentendo eventuali integrazioni documentali senza pregiudicare la validità delle stesse. fissare poi una data certa entro la quale erogare i rimborsi, evitando che chi abbia fatto ricorso al condono - ma questo l'ha chiarito anche il Sottosegretario - o a sanatorie fiscali

prima della vigenza del decreto possa determinare situazioni di illiceità. Questo provvedimento, signor Presidente, appare di corto respiro, opaco nella sostanza, confuso nelle modalità applicative. Esso costituisce una falsa soluzione che dimostra la reale volontà del Governo, anche attraverso il decreto-legge n. 262, di non dare corso alla sentenza europea; confermato dalla mancata abrogazione, in premessa, delle norme oggetto della censura comunitaria, accrescere vedo così l'indeterminatezza degli obiettivi dell'Esecutivo. Sono evidenti i rischi di tale intervento: di incorrere in una nuova censura da parte delle autorità comunitarie per violazione del principio di effettività delle pronunzie. Ciò rappresenterebbe una scelta grave e una lesione dei diritti dei contribuenti italiani. Sarebbero inevitabili nuovi ricorsi, nuove sentenze, nuove infrazioni, nuove pronunce e nuove condanne. Una questione di particolare delicatezza concerne la determinazione del periodo di imposta a partire dal quale può essere richiesto il rimborso dell'IVA indebitamente versato. Credo che occorrerebbe applicare il termine di decorrenza della prescrizione ordinaria e quindi fare riferimento ai pagamenti effettuati dal 1996 e non dal 2003.

di una sentenza della Corte di giustizia e quindi avessimo la possibilità di discutere nel merito della

riconosca il diritto al rimborso dell'IVA per l'acquisto di veicoli non afferenti l'attività produttiva dell'impresa

Perché di questo si tratta, non di una discussione generica sul diritto dei contribuenti ad ottenere tempestivamente il rimborso di quanto eventualmente pagato per tributi. Peraltro, se di questo si trattasse, credo che tutti avremmo la preoccupazione di far sì che questo rimborso avvenisse nei tempi più rapidi, nelle modalità più più accelerate possibili; cosa che sembra nella preoccupazione dei colleghi dell'opposizione che hanno parlato fino ad ora, magari dimenticando il fatto che solitamente il normale cittadino, che si è trovato a versare qualche euro o qualche migliaia di euro in più al fisco, deve poi aspettare tempi biblici per la restituzione. In questo caso vi è questa enorme preoccupazione affinché la restituzione avvenga nei tempi più rapidi possibili. Si parla addirittura di maltolto. Mi chiedo se può essere considerato maltolto da parte dello Stato a danno dei cittadini l'IVA che lo Stato ha incassato per l'acquisto da parte delle imprese di autoveicoli e per e per le spese di esercizio di questi autoveicoli, che non hanno afferenza con le attività che l'impresa svolge. Sostanzialmente, e per dirla brutalmente, è la pretesa, riconosciuta dalla Corte di giustizia, che l'IVA che le imprese scaricano per acquistare il mezzo di trasporto sportivo o il SUV o il fuoristrada per il rampollo dell'impresa debba essere restituita. Di questo si tratta: non è in discussione il diritto al rimborso dell'IVA per i camion, per le ruspe, per i veicoli di lavoro. Si tratta di veicoli non riferiti e non afferenti alle attività delle imprese. Se la inquadriamo in questi termini, credo che il nostro ragionamento dovrebbe essere comune e comunemente rivolto a considerare questa sentenza dalla Corte di giustizia non soltanto un atto cui rivolgerci con l'obbedienza, ma un atto che solleva e sollecita riflessioni. Peraltro, queste riflessioni non soltanto sono state sollecitate dalla stessa sentenza - lo ha ricordato il collega D'Amico ma queste riflessioni sono sollecitate da una persistenza di iniziativa della Commissione europea che chiede al Governo italiano di volta in volta di specificare quelle aree che possono essere sottratte alla norma del rimborso dell'IVA; cosa che i Governi che si sono succeduti, magari con tempestività non proprio commendevoli, hanno fatto nel corso degli anni; su cui a partire dal 2001 di fronte ad una precisa richiesta, sollecitazione e posizione della Comunità europea che chiede al Governo italiano di specificare, e una volta per tutte, le aree e le fattispecie per cui l'IVA non fosse rimborsabile, il Governo che ha governato nel nostro Paese è stato zitto! Da questo punto di vista ha ragione il collega D'Amico quando dice: nello stesso momento in cui approviamo questo decreto, il Governo si faccia carico di indagare circa le responsabilità di tanta grave omissione.

e che graverà per altri 13 miliardi e 400 milioni nei prossimi anni. Questo è il punto.

Confindustria, addirittura di furto a proposito dell'utilizzazione del TFR per investimenti pubblici. Vorrei chiedere se tanto zelo è messo dalla Confindustria nel sostenere una vertenza attivata da un'impresa che aderisce alla stessa, nella consapevolezza che si trattava di una materia così delicata e controversa. Tale semplicemente sull'interpretazione formale della norma, o sulla intempestività o sulla sordità o sulle omissioni e disattenzioni del Governo italiano nel marcare, appunto, questa prerogativa dello Stato di distinguere tra chi è titolare legittimo del diritto di rimborso dell'IVA e chi non lo è, in ragione di spese che non possono rientrare nella fattispecie di spese finalizzate allo sviluppo delle attività produttive. Di questo si tratta.

e mettendo in primo piano l'interesse collettivo dello Stato e della società italiana rispetto a quello del singolo, del singolo, mi sarei aspettato che si addivenisse non soltanto all'approvazione del decreto-legge come atto dovuto nei confronti della sentenza della Corte di giustizia delle ma anche come adesione a un criterio perfino pedagogico nei confronti dei comportamenti dei comportamenti delle imprese a proposito dell'acquisto di questi beni. Qualche collega in Commissione ha detto che, in fondo, si tratta del riconoscimento che

Francamente, mi sembra eccessivo che tale *benefit* sia messo a carico del contribuente del nostro Paese.

in Commissione e gli ordini del giorno di cui siamo anche cofirmatari. Ci auguriamo davvero che lo Stato italiano e questo Governo si mettano nella condizione di capire cosa è successo in passato e cosa ha determinato questa situazione e che, peraltro, si mettano strutturalmente nella condizione che quanto è accaduto non si ripeta.

Non posso che iniziare dal 14 settembre 2006, quando la Corte di giustizia delle Comunità europee, intervenendo in merito alla controversia tra la società Stradasfalti S.r.l. e l'Agenzia delle entrate sulle pretese di rimborso IVA che la società dichiarava di aver indebitamente versato dal 2000 al 2004 per l'acquisto, l'uso e la manutenzione di veicoli da turismo non rientranti nell'oggetto dell'attività propria della società, emetteva una sentenza favorevole alla società, imponendo, in conseguenza, il naturale adeguamento. Seguiva, quindi, il decreto-legge 15 settembre 2006, n. 258, di cui oggi il Governo chiede la conversione con il disegno di legge Atto Senato n.

cui interno non potrebbero essere ravvisate responsabilità da parte dell'attuale Esecutivo. Questo Governo è riuscito invece nell'ardua impresa di inanellare una serie impressionante di errori, i cui effetti negativi speriamo non vengano a ricadere nei prossimi mesi sugli incolpevoli contribuenti. Innanzitutto, come si fa a definire tale provvedimento come atto di esclusiva natura procedimentale che non interviene sulla disciplina sostanziale della detraibilità dell'IVA, non determinando così la presenza di oneri finanziari? Certo, se se ne dà un'interpretazione letterale, è chiaro che il provvedimento si riferisce solo alle procedure e alle modalità di rimborso; ma è qui il vostro gravissimo errore, frutto non so dire se di colpa o di dolo. Il nostro parere è che sarebbe stato assolutamente necessario cogliere la presente opportunità per dar vita a un provvedimento di ampio respiro, capace di affrontare la revisione della normativa IVA, sia al fine di dare certezza ai contribuenti, sia al fine di evitare salti nel buio per i conti pubblici. Al contrario, voi avete fatto respirare un'aria di incertezza sulla quantificazione del rimborso (ancora oggi non sappiamo - ma, soprattutto, non sapete - a quanto ammonterebbe) facendo alternare cifre, tutte considerevoli, in verità, ma altrettanto considerevolmente distanti tra loro in termini quantitativi. Sono o non sono 15 miliardi di euro? Credo che il Governo debba finalmente dire una parola chiara Il problema, peraltro, a tale riguardo, è duplice: da un lato, vi è la dimostrazione che l'attuale Esecutivo non è in grado di conoscere e quindi di valutare le varie poste che potrebbero incidere sui conti pubblici; dall'altro, vi è la preoccupazione sul tipo di copertura che intende dare al provvedimento che, sulla base dei primi segnali, non potranno che abbattersi sui soggetti più deboli. A tal riguardo, quando chiedevamo di discutere congiuntamente della parte del decreto fiscale dov'è prevista la compensazione e la copertura di questo provvedimento, non lo facevamo a caso, ma perché avvertivamo il bisogno che su questo argomento ci fosse una coerenza di fondo che garantisca il contribuente e soprattutto le imprese. Siamo critici anche in merito alla procedura. Nonostante la Corte di giustizia delle Comunità europee in più occasioni si sia espressa contro l'introduzione di limiti e di orpelli nell'applicazione delle proprie sentenze ed abbia censurato qualsiasi atto, fatto o procedura che ne potesse inficiare il principio di effettività, avete insistito sull'utilizzo della procedura telematica, denotando una preoccupante propensione a concezioni dirigistiche anche nelle questioni più praticamente operative. non solamente volete far valere i vostri criteri nell'adozione di questo provvedimento, ma pretendete anche di dire come e in che misura si debbano muovere i cittadini contribuenti per poter affermare e riaffermare un loro diritto. Il nostro parere - lo dicevo prima - è che sareste dovuti intervenire contemporaneamente all'individuazione delle procedure di rimborso con l'abrogazione delle norme superate dalla sentenza della Corte di giustizia, anche al fine di evitare pericolosissimi vuoti normativi, e con la ricerca di misure necessarie a coprire strutturalmente e non temporaneamente tali costi. Avreste dovuto farlo con un ampio e articolato dibattito, anche perché la scopertura attuale equivale ad una minifinanziaria che è sotto gli occhi di tutti e rappresenta un problema per tutti. Invece, l'impressione è che ancora una volta l'onere si abbatterà sul sistema delle imprese in misura addirittura superiore ai presunti benefici «presunti») che vorreste accreditare con il cosiddetto cuneo fiscale inserito nel disegno di legge finanziaria. Tutto ciò non è avvenuto, in aperto dispregio delle regole più elementari di democrazia, violando i princìpi generali dello statuto del contribuente, motivo per cui non è irrealistico pensare ad una serie infinita di ricorsi e di provvedimenti di salvaguardia da parte delle categorie colpite. Peraltro, con il taglio politico che avete voluto dare avete poi inferto un duro colpo ad un altro principio cardine del sistema tributario, la certezza del contribuente. Navigate a vista, e lo sappiamo, ma questo è un lusso che possiamo consentire a voi perché siamo convinti che vi porterà fuori rotta, non possiamo permettere che l'incertezza possa costituire la regola nella programmazione delle imprese. Un'impresa, grande o piccola che sia, sia sottoforma individuale che societaria, e anche al di là della propria caratterizzazione giuridica, ha bisogno di avere di fronte un quadro normativo, anche in materia tributaria, certo e di medio-lungo periodo per poter programmare la propria attività. I primi atti dell'attuale Governo non vanno in questa direzione, tutt'altro. è un esempio la vostra ostilità a considerare qualsiasi ipotesi di compensazione o di detrazione. Ci volete spiegare perché? Lo abbiamo chiesto anche in sede di Commissione finanze; abbiamo chiesto quale fosse la *ratio* che sottosta a questo tipo di provvedimento, soprattutto a questo tipo di atteggiamento, un atteggiamento di chiusura assolutamente incomprensibile,

e siete condannati vita natural durante a venire qui, in quest'Aula senza un adeguato provvedimento del relatore. Allora perché? Forse perché la detrazione e la compensazione sono immediatamente attivabili dal contribuente, mentre il rimborso segue procedure diverse? Se è così, il Governo ha il dovere di dirlo nella sede deputata, cioè in Parlamento, in quest'Aula, nel Senato della Repubblica. Ma se è così, il Governo deve pure ammettere che i tempi di effettivo rimborso non sono assolutamente certi, violando in tal modo il già richiamato principio di effettività, ribadito in più circostanze dalla Corte di giustizia e richiamato dai colleghi intervenuti poco fa nell'esame di questo provvedimento. Colleghi, credo o, almeno, mi auguro di aver sinteticamente rappresentato i motivi per i quali Alleanza Nazionale ha espresso critiche e rilievi al provvedimento. Ci siamo soffermati su questioni puramente tecniche, ma ci sono altre questioni di natura squisitamente politica. Pur in presenza di un provvedimento che avrebbe potuto trovare consensi in ampia parte dello schieramento politico presente in questo ramo del Parlamento, il Governo si è chiuso in un'incomprensibile refrattarietà a recepire i suggerimenti e le proposte migliorative che Alleanza Nazionale e il centro‑destra hanno ritenuto di proporre. Non so dire se si sia trattato di presunzione oppure di arroganza; di certo, non è parsa questa una dimostrazione di forza, semmai è stata una dimostrazione di debolezza, peraltro non molto abilmente dissimulata. Per quanto riguarda Alleanza Nazionale, intendiamo far emergere tutte le vostre debolezze, tutte le vostre carenze, tutti i vostri limiti, le vostre incoerenze, le contraddizioni, in maniera sicuramente e politicamente composta, consapevoli della caduta verticale di credibilità che siete stati superbamente capaci di realizzare in pochissimi mesi. Signor Presidente, onorevoli colleghi, esame è un provvedimento, per dir così, di natura funzionale, nel senso che, non essendo data al Parlamento discrezionalità di sorta per la costruzione e il modellamento dello stesso, ma dovendo soltanto dare esecuzione ad un provvedimento giurisdizionale, qual è quello della Corte di giustizia europea, avrebbe dovuto essere tale da non destare divisioni, né contrapposte posizioni tra maggioranza e opposizione. Così non è stato, per i seguenti motivi. Si è voluto, da parte della maggioranza, non dare la certezza del diritto a chi va a credito in forza di un provvedimento giurisdizionale. E non giova, in questa sede, ripercorrere l'*iter* del provvedimento della Corte di giustizia, dal momento che ognuno deve fare il proprio mestiere, o dico meglio, ognuno deve assolvere alla sua funzione istituzionale. In questa sede non si può recriminare sulla decisione della Corte di giustizia: il giudicato è un giudicato e una sentenza è una sentenza. Le sentenze, per esigenze anche di natura pedagogica, le istituzioni debbono rispettarle: guai se all'opinione pubblica diamo ad intendere che una sentenza può essere disattesa o raggirata! E nel caso di specie, di fatto, la si raggira. La si raggira nel momento in cui si pone un termine molto più breve di quello che è dato allo Stato per accertare l'imposta e pretenderne la riscossione, fissando al 15 dicembre il termine entro il quale agire per via telematica. Non tutti ancora usano lo strumento telematico in Italia, nonostante ogni migliore sforzo applicato dal Governo Berlusconi per perseguire l'informatizzazione del Paese - il tempo che abbiamo avuto è stato breve - e pertanto dire «per quella via ed entro il 15 dicembre devi chiedere qual è il tuo credito per poter accendere il tuo diritto»

allo Stato per poter accertare l'eventuale omesso versamento da parte del cittadino, per un'esigenza di equilibrio postulata dallo Statuto dei diritti del contribuente. Fui presentatore di uno dei disegni di legge in di maggio, cui seguì quello del Governo, di settembre. Ma non voglio rivendicarne la primogenitura: la primogenitura è del Parlamento, che ha voluto lo Statuto dei diritti per dare al cittadino italiano la possibilità di essere considerato tale e all'Erario di essere qualificato pubblica amministrazione, ponendo le parti in posizione paritetica. qualcosa di più grave, nel momento in cui non si stabilisce il termine entro il quale la pubblica amministrazione assume l'impegno al rimborso. Che sia chiaro: avete tutta la nostra comprensione. Potrà essere un termine lungo, ma va fissato. In assenza di un termine, il diritto non è perfetto: al cittadino creditore, per esempio, non è data la facoltà di cedere il credito, perché nessuno accetta la cessione di un credito, come è giusto che accada quando si è creditori, in mancanza di un termine

di avere un diritto compiuto, qual è quello di un credito, che tra gli elementi essenziali postulati dal codice civile ha il termine per l'esecuzione dell'obbligazione, vi preghiamo di compiere tutti gli adempimenti che un'amministrazione pubblica, che abbiamo l'obbligo di rispettare anche quando è governata da qualcuno che non condivide le nostre tesi politiche, può adempiere. Proprio per un'esigenza di natura pedagogica, amici che avete parlato di pedagogia, che esempio diamo

il molto rispettabile, e che non sono degno di menzionare, San Giuseppe da Copertino, che volava? Gli imprenditori non volano, i professionisti non volano, dategli il credito che essi vantano. il decreto al nostro esame assume grande rilievo poiché si propone, com'è noto, di regolare il rapporto tributario tra una moltitudine di contribuenti, esercenti attività di impresa e professionisti, e l'erario, a seguito della nota pronuncia della Corte di giustizia delle Comunità europee in materia di detraibilità dell'IVA pagata dai predetti soggetti per l'acquisto di autovetture e veicoli in genere. Se non fosse per l'enorme rilevanza dell'ammontare del debito erariale scaturito dall'accertamento giudiziale suddetto e se il contenuto del decreto non ponesse complessi problemi afferenti alla gestione del bilancio dello Stato, il provvedimento non meriterebbe estesi ed approfonditi commenti e valutazioni. Infatti, il decreto che siamo chiamati a convertire in legge si limita a regolare le modalità attraverso le quali rendere certi e liquidi i crediti dei contribuenti, a fissare un termine per la presentazione delle domande, a vietare compensazioni tra il credito pregresso e i debiti di imposta correnti, in tal modo affermando certezze a favore ed a carico delle imprese, dei professionisti e dello Stato. In realtà, dietro il dato contenutistico del provvedimento, relativamente semplice, si nascondono le suindicate complesse problematiche, che è il caso di evidenziare in questo dibattito, come già si è cercato di fare sia nella Commissione di merito che nella Commissione bilancio. Innanzi tutto, credo meriti apprezzamento la tempestività con la quale il Governo ha inteso regolare la vicenda che è venuta a determinarsi nel modo predetto. Seppure sospinto dall'esigenza di evitare effetti dirompenti sulla finanza pubblica e possibili abusi derivanti dalla teorica possibilità di compensazione da parte dei contribuenti, l'intervento del Governo va sottolineato proprio perché esso è idoneo a definire i rapporti sorti antecedentemente alla sentenza, fissando tempi e procedure di riconoscimento dei crediti. Altra cosa è la liquidazione, sulla quale si dovrà successivamente intervenire.

ma è altrettanto vero che dette sentenze non attribuiscono al cittadino l'automatica possibilità di ritenersi titolare di un diritto certo ed immediatamente esigibile, bensì legittimano gli stessi ad azionare la pretesa avanti al giudice italiano, che dovrà nel caso anche procedere all'accertamento della situazione sostanziale sottostante. Ecco quindi che l'aver disposto una procedura ricognitiva del diritto non soltanto ha evitato immediati e negativi effetti sul bilancio dello Stato, ma ha anche permesso e permetterà ai numerosissimi contribuenti interessati di ottenere il rimborso, in moneta o mediante futura compensazione, senza essere costretti ad attivare una procedura giudiziaria. Si è prodotto dunque un ampliamento, ovvero un giusto riconoscimento e non un restringimento, come è stato sostenuto, dell'interesse dei diritti dei contribuenti, i quali potranno ottenere in via amministrativa e senza dispendio di energie, di tempo e di denaro ciò che avrebbero potuto pretendere soltanto in sede giudiziaria. In secondo luogo, è senz'altro utile rilevare che il Governo e il Parlamento stanno facendo buon uso del loro potere di legiferare anche relativamente alla corretta appostazione in bilancio dell'onere finanziario scaturito dalla sentenza di cui ci stiamo occupando. È stato sostenuto e contestato da parte dei colleghi dell'opposizione che il Governo prima e il Parlamento dopo avrebbero dovuto individuare immediatamente una fonte di copertura dell'onere finanziario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e della legge di contabilità; così non è per le ragioni che abbiamo già sostenuto in Commissione bilancio e che qui è il caso di riaffermare Ipotesi come quella di cui ci stiamo occupando sono esattamente previste e disciplinate dalla legge di contabilità, che al comma 7 dell'articolo 11-*ter* prevede, appunto, che nel caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali, recanti interpretazioni della normativa vigente, suscettibili di determinare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Parlamento con propria relazione e assume le conseguenti iniziative legislative. Si badi che detta procedura esclude l'obbligo di prevedere apposita copertura finanziaria, siccome i diritti che generano oneri a carico del bilancio dello Stato, accertati in sede interpretativa, giudiziale, devono ritenersi già riconosciuti dall'ordinamento e quindi non necessitano dell'emanazione di norme positive, attributive del diritto medesimo, nel quale caso, sì, occorrerebbe individuare la copertura, seguendo il normale *iter* di formazione delle leggi. La *ratio* di tale norma di contabilità è evidente: il Governo e il Parlamento non possono rincorrere la giurisprudenza ogni volta che questa emani pronunce interpretative su norme generatrici di oneri a carico del bilancio dello Stato. Si determinerebbero, in tal caso, conseguenze aberranti e incidenti anche sull'autonomia costituzionale del Parlamento. Allora, bene ha fatto il Governo a seguire la procedura disciplinata con il decreto; bene ha fatto a comunicare al Parlamento gli effetti finanziari della sentenza della Corte di giustizia nella sede propria, cioè con la Nota di aggiornamento al DPEF. Con essa, infatti, si è correttamente reso edotto il Parlamento dell'impatto finanziario della vicenda di cui ci stiamo occupando, stimato in 3,7 miliardi di euro per il 2006, e, in ragione della competenza economica, maggiori oneri stimati in 13,4 miliardi di euro, per il pagamento degli arretrati relativi agli anni dal 2003 al 2005. Tale ingente onere ha effetti - e non potrebbe essere altrimenti - sull'indebitamento netto, che in tal modo viene a collocarsi al 4,8 per cento del PIL, con un aggravio rispetto alla precedente stima dell'1,2 Di quale trucco contabile si tratti - come affermato anche oggi dal senatore Baldassarri nella discussione sulla Nota di aggiornamento al DPEF - non è dato Si riconosce un diritto e i termini dei rimborsi non potranno che essere successivamente fissati, anche in ragione dell'esatta quantificazione dell'onere che scaturirà dalle domande dalle domande che saranno presentate dai contribuenti; si disciplinano le modalità di presentazione delle istanze; si rileva l'impatto sul debito pubblico. Non si vede cos'altro il Governo avrebbe dovuto fare e non ha fatto. Piuttosto, le attuali opposizioni dovrebbero spiegarci perché il Governo Berlusconi non ha inteso mantenere l'impegno, che fu assunto in sede comunitaria nel 2000, di riesaminare la misura limitativa di cui stiamo discutendo a partire dall'anno 2001, modificando il regime restrittivo del diritto alla detrazione dell'IVA, per troppo tempo prorogato. Anche questa, signori dell'opposizione, è dunque un'eredità del vostro Governo, che avrebbe potuto e dovuto attivarsi in sede comunitaria negli ultimi cinque anni, per modificare la norma in questione. Per queste ragioni sosteniamo convintamente questo decreto, che ci auguriamo possa essere ulteriormente

provenienti dalle opposizioni, per esempio differendo ulteriormente il termine per la presentazione delle domande e in ogni caso non sopprimendo il diritto dei contribuenti ad ottenere il rimborso anche dopo la scadenza di detto termine, alle condizioni indicate nell'emendamento medesimo. Si potrebbe opinare - e ciò è legittimo sulla congruità, sull'adeguatezza delle regole di bilancio di cui ho sopra sinteticamente parlato, di fronte a casi come quello di cui ci stiamo occupando. Ciò, però, appartiene ad uno spazio di dibattito politico che possiamo aprire, ma che dovrebbe necessariamente sfociare in una modifica della legge di contabilità. Oggi il sistema è quello che ho sinteticamente richiamato ed al quale dobbiamo necessariamente attenerci. Anche in passato la procedura seguita è stata la stessa. Richiamo, per esempio, la vicenda della tassa sulle società, numerose altre pronunce in materia previdenziale ed altro. Oggi non possiamo che attenerci alla norma richiamata e alla prassi parlamentare in passato Non possiamo che ribadire il nostro sostegno convinto a questa iniziativa legislativa, che introduce chiarezza e certezza nel rapporto tra contribuenti e amministrazione finanziaria, che recepisce una statuizione del massimo organo di giustizia comunitario e che registra l'impatto sull'indebitamento dello Stato, peggiorato non certo per responsabilità di questo Governo e di questa maggioranza che, anzi, si sono immediatamente attivati anche con la finanziaria e il decreto-legge in materia fiscale ad essa collegato per porre rimedio

sulle dimissioni reiterate dai senatori Malabarba e Turco. La seduta potrà pertanto proseguire oltre l'orario già stabilito. Comunico inoltre che, sempre all'unanimità dei Capigruppo, sono stati riassegnati in sede deliberante alle competenti Commissioni il disegno di legge recante istituzione di una Commissione d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti, nonché i documenti relativi alle inchieste monocamerali sugli infortuni sul lavoro e sull'uranio impoverito, già all'ordine del giorno dell'Assemblea. Le Commissioni 13a, 11a e 4a, rispettivamente competenti per l'esame di tali provvedimenti, sono pertanto autorizzate fin d'ora a convocarsi. Ricordo che domani mattina saranno poste all'ordine del giorno le mozioni sulle vicende connesse al discorso tenuto da Papa Benedetto XVI a Ratisbona. Come già comunicato per le vie brevi ai Gruppi, la Presidenza, ai fini di una migliore organizzazione del dibattito, ha ripartito i tempi degli interventi nella misura di 20 minuti a Gruppo, comprensivi di illustrazione, discussione generale e dichiarazioni di voto. Sempre domani mattina, a conclusione di tale dibattito, inizierà l'esame del decreto-legge sulla missione in Libano, per il quale sono stati ripartiti i tempi tra i Gruppi. Domani pomeriggio il *question time* riguarderà la vicenda della bambina bielorussa ospite di una famiglia genovese. Ulteriori comunicazioni sul calendario dei lavori, approvato all'unanimità dalla Conferenza dei Capigruppo, saranno rese all'Assemblea nel corso della seduta antimeridiana di domani.

oltre un punto percentuale di PIL, cioè gran parte della manovra finanziaria, se non fosse intervenuto questo decreto per cercare di identificare un modo per risolvere problemi del passato e poi naturalmente gettare le basi per affrontare il tema del futuro. Com'è stato ricordato, ci riferiamo ad una sentenza che, sulla base della protesta di una ditta di costruzioni, ha contestato l'applicazione di un norma italiana in contrasto con la sesta direttiva comunitaria; già nel 2001 fu introdotta una variazione consentendo la detrazione al 10 poi però vi è stato un periodo lungo durante il quale è intervenuta la contestazione della ditta, le sentenze prima del giudizio tributario, poi l'appello a Bruxelles, senza che intervenisse una efficace controffensiva del Governo. quali sono gli argomenti del Governo: rispondo che sono quelli del Governo che c'era nel momento in cui c'era la procedura di fronte alla Corte di giustizia europea, cioè il Governo precedente. Non c'è dubbio che c'è stata una debolezza nell'affrontare con provvedimenti adeguati i problemi che questa sentenza avrebbe probabilmente posto, né è bastato portare dal 10 al 15 per cento nell'anno vigente la possibilità di detrazione, perché la sentenza della Corte è una sentenza in sostanza, dice ad ogni piè sospinto che il problema di fondo è la mancata consultazione, prevista dalla direttiva, del comitato che deve autorizzare le legislazioni nazionali in materia. Il fatto di non avere innovato dal punto di vista legislativo, limitandosi a dei ritocchi percentuali sulle detrazioni, ha creato il problema che noi oggi dobbiamo affrontare. Il decreto ha bloccato non solo la possibilità di compensare fino al 15 dicembre, ma ha anche evitato che il contribuente potesse compensare, nell'incertezza di dovere poi restituire, cioè ha cercato di fare chiarezza. È intervenuta nella discussione la richiesta di avere più tempo, di poter consentire che lo Statuto del contribuente non venisse contraddetto, i famosi sessanta giorni almeno tra il momento in cui il direttore dell'Agenzia delle entrate produrrà la certificazione necessaria e il momento in cui dovrà essere presentata la domanda: questo è oggi risolto a prima firma della senatrice Thaler Ausserhofer, che avrebbe dovuto essere relatrice di questo provvedimento, emendamento che il Governo condivide e accoglie e che secondo noi risolve positivamente il problema portando al 15 aprile 2007 la possibilità di presentare le domande per via telematica, non di produrre la documentazione, che verrà eventualmente successivamente richiesta dagli uffici (deve quindi essere conservata ma non obbligatoriamente presentata per via telematica entro il 15 aprile), introducendo un periodo più lungo, di conseguenza, per la decadenza, come del resto c'è stato suggerito dalla Commissione dell'Unione Europea. Si tratta quindi già oggi, con l'emendamento 1.100, che io considero parte integrante del testo del decreto, una possibilità di svolgere le cose in modo che i contribuenti abbiano la certezza di ciò che faranno in futuro e di affrontare correttamente anche la prospettiva. Nell'emendamento 1.100 c'è un altro dato che il Governo condivide e riguarda la procedura con cui intervenire se vi sarà, da parte dell'Unione Europea, il consenso ad un'ipotesi che abbiamo

sulla base dell'applicazione individuale del principio dell'inerenza, cioè precisando quanta parte di queste auto sia effettivamente per uso aziendale, in modo tale che questo principio possa consentire

che preferisca andare ad una transazione bonaria con l'amministrazione fiscale, la possibilità di forfetizzare questo rimborso. L'ipotesi è quella di una forfetizzazione per settori di attività; è possibile ricostruirla con gli studi di settore e in questo modo l'applicazione diventerebbe per tutti estremamente semplice. In sostanza, l'emendamento 1.100 che, ripeto, il Governo condivide integralmente, consente di avere l'immediata applicabilità di un consenso dell'Unione Europea, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*, ad un meccanismo di doppio binario: o l'analitico con inerenza oppure la possibilità di avere una forfetizzazione. C'è naturalmente anche il futuro e il futuro trova una sua applicazione già oggi nell'ambito di un combinato disposto della norma che l'emendamento 1.100 propone e di quanto prevede il decreto fiscale in vigore, oggi in esame alla Camera. Per il futuro occorre avere le risorse; per avere le risorse e non incidere sui saldi di finanza pubblica, il Governo ha proposto di intervenire su un sistema di imposte dirette per l'impresa, che sono di libera determinazione del Parlamento italiano.

Tale possibilità è, quindi, oggi integralmente coperta dalle norme già individuate, mentre il pregresso è coperto dalla tabella A della legge finanziaria in esame alla Camera, che prevede una regolazione per debito pregresso e quindi in tabella A vengono previste le risorse necessarie per pagare quanto si è determinato fino ad oggi come credito dei contribuenti. Questo per dire che il decreto, con le modifiche dell'emendamento 1.100, che il Governo condivide, consente di avere già tutta la procedura per il futuro. Con i due provvedimenti, legge finanziaria e decreto, si finanzia sia la regolazione debitoria pregressa sia il futuro e di conseguenza a noi sembra sia completamente assolto il compito di far fronte alla sentenza comunitaria. Non condivido i profeti di sventura che anche in quest'Aula hanno detto che ciò genererà ulteriori contenziosi: no, in questo modo si va a sistemare una partita molto impegnativa che, se non affrontata, avrebbe creato un problema enorme per i saldi di finanza pubblica e praticamente riscritto la finanziaria di quest'anno e anche degli anni futuri. futuri. A questo punto possiamo dire che c'è il pieno rispetto della sentenza e che viene rispettato lo Statuto dei diritti del contribuente, su cui c'è stata tanta insistenza anche nei lavori di Commissione.

parere non ostativo». «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta osservando quanto segue: la sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 14 settembre 2006 rientra nelle fattispecie disciplinate dall'articolo 11-*ter*, comma 7, della legge n. 468 del 1978, secondo cui il Governo - a fronte di andamenti di finanza pubblica divergenti dalle previsioni - riferisce al Parlamento con propria relazione assumendo le conseguenti iniziative legislative, esigenza in parte soddisfatta, sul piano sostanziale, dalle indicazioni fornite nella nota di aggiornamento al Documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 2007-2011; fermi restando gli attuali criteri di verifica del rispetto dell'articolo 81, comma 4, della Costituzione, risulterebbe inoltre utile che il Governo, in sede di relazioni tecniche sui provvedimenti di spesa, indicasse - a fini informativi e di documentazione - l'impatto della innovazione normativa su ciascuno dei saldi di finanza pubblica (saldo netto da finanziare del bilancio statale, fabbisogno e indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni)». esame e sugli emendamenti. parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 01.1, 1.33, 1.34, 1.35, 1.37, 1.19, 1.21, 1.27, 1.28, 1.29, 1.30 e 1.36. Esprime altresì parere contrario sugli emendamenti 1.23, 1.24, 1.25 e 1.26. Con riferimento all'emendamento 1.100, esprime parere di nulla osta sulla lettera *a)*, parere contrario sulla lettera *b)* e parere di nulla osta sulla lettera osservando tuttavia che apparirebbe ragionevole collocare la disciplina ivi contenuta nel medesimo provvedimento volto a disciplinare interamente la materia. Esprime quindi parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sui subemendamenti 1.100/1, 1.100/2, 1.100/3 e 1.100/4. Esprime infine parere di nulla osta su tutti i restanti emendamenti».

prima di illustrare l'emendamento 1.100, mi preme formulare una raccomandazione generale al Governo, ossia quella che, nel formulare testi normativi in materia fiscale e tributaria, si dovrebbero tenere ben presenti i princìpi stabiliti dallo Statuto dei diritti del contribuente; princìpi importantissimi che tutti gli schieramenti politici hanno voluto e appoggiato fortemente. Con l'emendamento proposto vengono modificate alcune disposizioni del testo del provvedimento presentato dal Governo, proprio in virtù dei princìpi previsti dallo Statuto, e soprattutto si intende rendere più esplicite e puntuali alcune disposizioni affinché su di esse siano limitate al massimo possibili interpretazioni diverse. Al punto 1 della lettera *a)* si precisa che i soggetti passivi destinatari della normativa sono quelli che hanno effettuato nell'esercizio dell'impresa, arte o professione acquisti e importazioni

si inserisce una disposizione di proroga dei termini per presentare la richiesta di rimborso: dal 15 dicembre 2006 al 15 aprile 2007. Si propone, poi, di eliminare le parole: «a pena di decadenza», per dare la possibilità a tutti i soggetti interessati di presentare le istanze anche dopo il 15 aprile 2007. Ritengo necessarie queste due modifiche, perché in linea con i principi dello statuto del contribuente. Da una parte, la proroga lascerebbe un tempo congruo ai contribuenti per aderire agli obblighi imposti dall'amministrazione finanziaria, dall'altra, darebbe la possibilità di non perdere il diritto al rimborso se l'istanza non venisse presentata entro il 15 aprile.

Viene infatti prevista la facoltà di scegliere tra una richiesta di rimborso in misura forfetaria e una di rimborso integrale di quanto indebitamente versato. Nel primo caso si farà riferimento alle prescrizioni di un regolamento attuativo redatto anche in base alle percentuali di utilizzo della detraibilità dell'IVA differenziata per settori, in accordo con l'Unione Europea.

La maggioranza tardivamente si è resa conto che i termini del 15 dicembre erano troppo ravvicinati per cui

apprezzato. Noi non apprezziamo la seconda parte dell'emendamento, laddove introduce criteri di forfetizzazione: come dire al contribuente di accontentarsi di poco

e 2005, si ha una smentita di quello che ha dichiarato il Governo sul fatto che per la copertura di 13,4 miliardi di euro - ripeto, signori della maggioranza e dell'opposizione, 13,4 miliardi di euro - ancora non sono stati emessi i BOT, BOT, di cui si ha notizia nella relazione di accompagnamento alle dichiarazioni che il sottosegretario Casula ha dato sulla Nota di aggiornamento del DPEF. Pertanto, a questo punto si ha una triangolazione

di un ammuino tra dei decreti-legge e una finanziaria che costituiscono la negazione di quello che dovrebbe essere il rigore richiamato solo a parole nel Documento di programmazione economico-finanziaria e che qui viene negato per dichiarazione dello stesso Governo. Pertanto, siamo contrari all'emendamento

determinata con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Ma come? È il direttore dell'Agenzia delle entrate che decide la forfetizzazione di un importo che deve essere restituito a un imprenditore a seguito della nota sentenza europea? Dovremmo - noi lo avevamo proposto a livello emendativo - perlomeno

chiarire con la dovuta pacatezza al senatore Ferrara che, per ciò che riguarda la regolazione debitoria - formula che ha un'influenza sulla finanza pubblica c'è un accantonamento in tabella *a)* della legge finanziaria (che, del resto, potete tranquillamente controllare) di 3 miliardi per gli anni Se la regolazione debitoria si dovesse rilevare insufficiente (in sostanza questo è debito), ci sarà un'integrazione per la parte che dovesse essere insufficiente,

ci sono le entrate sufficienti per coprire la previsione di spesa. Quindi, i conti sono del tutto chiari e in ordine: regolazione debitoria per il passato, con l'accordo dell'Unione Europea,

che c'è stato soltanto un condono, quello del 2002. Ha quindi sconfessato l'idea che sia stato approvato un condono l'anno da parte del precedente Governo, mentre abbiamo scoperto che questa legge finanziaria presenta un condono previdenziale, cosa che era stata sempre negata.

abbiamo raggiunto l'accordo che alle ore 13 avremmo votato sulle dimissioni. Se ci fossero dichiarazioni di voto sul punto, credo sarebbe il caso di affrontare

Presidente, mi sembra di aver capito che stiamo per passare alla votazione sulle dimissioni del senatore Malabarba.

la finalità del decreto-legge n. 258 è quella di offrire una tutela concreta agli interessi di una larga fascia di contribuenti che hanno subito una limitazione alla detraibilità dell'IVA, limitazione ritenuta dalla Corte di giustizia delle Comunità europee contrastante con i princìpi comunitari in materia. Dunque, è impellente la necessità di procedere alla sua immediata conversione. Tale conversione consentirà di ottemperare proprio al dispositivo della sentenza emessa in data 14 settembre 2006, nella quale la Corte di giustizia ha osservato che gli Stati membri sono tenuti a conformarsi a tutte le disposizioni contenute nella 6a direttiva sull'IVA ed, in particolare, a quelle relative all'articolo 17, n. 7, primo periodo, che regolano le esclusioni dal regime delle detrazioni compatibili col principio del diritto alla detrazione. L'organismo giurisdizionale ha ritenuto incompatibile rispetto ai suddetti articoli la normativa italiana, che aveva introdotto una limitazione alla detraibilità detraibilità delle somme versate a titolo di imposta sul valore aggiunto negli anni 2002-2004 per l'acquisto, l'uso e la manutenzione di veicoli non rientranti nell'oggetto tipico dell'attività d'impresa. Dunque, per effetto della sentenza in questione, resa operativa proprio tramite le norme del decreto-legge al nostro esame, l'IVA sostenuta sulle suddette spese è ritenuta detraibile, qualora sussistano i requisiti dell'inerenza della spesa a operazioni imponibili e dell'afferenza all'esercizio dell'attività d'impresa. Per questa ragione il Governo ha opportunamente individuato una procedura per offrire una risposta certa ed immediata a quei contribuenti che hanno versato al fisco somme non dovute predisponendo un modello di richiesta di rimborso dei versamenti IVA non detratti. Da segnalare lo sforzo compiuto in Commissione bilancio dalla relatrice e dal rappresentante del Governo, sforzo purtroppo non andato a buon fine, di apportare modifiche migliorative al testo del decreto-legge con particolare riferimento alle modalità ed ai termini di esercizio del rimborso, sempre con l'obiettivo fondamentale di dare maggiore certezza ai rapporti tra cittadino e fìsco e di fornire adeguata risposta alle esigenze concrete fatte presenti dai contribuenti stessi. Proprio perché utili al conseguimento di tale obiettivo, accogliamo con particolare favore l'approvazione dell'emendamento 1.100 della senatrice Thaler Ausserhofer. Nell'auspicio che si possa arrivare a breve ad una complessiva revisione del regime di detraibilità dell'IVA, come auspicato da tutte le forze politiche, annuncio a nome dei Popolari-Udeur il voto favorevole al provvedimento in esame. *(Applausi

non adempia alle disposizioni della Corte di giustizia europea, ma si ponga anche in ulteriore contrasto con le stesse normative comunitarie in materia di IVA.

prospettiva originaria avrebbe dovuto dare giusta risposta alle aspettative dei contribuenti. Mi spiace che la discussione generale,

Signor Presidente, il mio intervento sarà molto breve. Annuncio il voto contrario di Alleanza Nazionale su un provvedimento congegnato e predisposto dal Governo, ulteriormente peggiorato dall'emendamento 1.100, presentato dalla senatrice Thaler e da altri esponenti del centro-sinistra, per aggirare e non applicare una sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee che era chiarissima nel suo contenuto. Con le modifiche testé introdotte con l'approvazione della seconda parte dell'emendamento della senatrice Thaler ed altri si rende assolutamente incerto il diritto al rimborso dei contribuenti in relazione sia

una buona occasione per rendere giustizia ai contribuenti che sono stati costretti negli anni a pagare somme molto ingenti e non dovute. Ancora una volta, purtroppo, dobbiamo votare contro perché si tratta di un vero e proprio imbroglio a danno dei contribuenti.

Presidente, ci troviamo a votare la richiesta di dimissioni di due colleghi. Non è la prima volta; in una precedente occasione, in dichiarazione di voto, mi sono permesso di notare che non per caso che il voto in queste circostanze è obbligatoriamente segreto.

Tuttavia, credo che una considerazione vada fatta e debba rimanere agli atti. Queste dimissioni, che ci vengono a più riprese sottoposte, hanno caratteristiche differenti: in alcuni casi, esse provengono da nostri colleghi che, per scelta personale, per circostanze sopravvenute, chiedono di potersi dimettere. In altri, queste dimissioni sono invece di rappresentanti del Governo che, evidentemente, ritengono

perché ritengo molto grave poter risolvere in questo modo un problema di ordine istituzionale e costituzionale che ha una sua grande rilevanza: quella del rapporto tra i poteri; il rapporto che deve vigere tra il Parlamento e l'Esecutivo. Su questo punto specifico, quello della separazione o meno dei poteri, e, in particolare, sulla possibilità o meno che membri del Governo possano anche sedere in Parlamento, molti dei colleghi presenti in quest'Aula sanno perfettamente che si giocò una partita importantissima in occasione dei lavori preparatori che poi portarono alla Costituzione della quinta Repubblica francese. Quel sistema viene anche chiamato sistema semi-parlamentare, chiamato sistema semi-parlamentare, proprio perché una delle sue caratteristiche è la divisione dei poteri che si è stabilita attraverso la statuizione dell'impossibilità per membri del Governo di essere contemporaneamente parlamentari. Si tratta di una scelta di grande momento nella storia del costituzionalismo europeo; non a caso, poi, a quell'occasione fecero riferimento tanti altri lavori preparatori quando dette giovani democrazie, che si inauguravano dopo la caduta del muro di Berlino, ebbero il problema di darsi delle Costituzioni democratiche. Non vorrei che questa scelta che, ripeto, è di grande delicatezza e che può essere risolto in un modo o nell'altro (vi sono motivazioni di di tecnica parlamentare, oltre che di ordine istituzionale che possono andare in un senso o nell'altro), venga da noi

il Parlamento e, per evitarlo, credo sia lecito da parte nostra chiedere delle assicurazioni esplicite e, cioè, che queste dimissioni non rappresenti un precedente che di fatto venga a fissare una incompatibilità che

Signor Presidente, onorevoli colleghi,

ma un'inopportuna elegia, un necrologio stile Terza internazionale, Politburo, del tra l'altro ottimo Capogruppo di Rifondazione, mi fece cambiare idea. Oggi però ci ritroviamo di fronte a queste dimissioni e voterò sì - il nostro Gruppo voterà sì - perché vi è anche un diritto alle dimissioni. Vorrei approfittare di questi brevi momenti per chiedere anche alla minoranza di valutare attentamente questa richiesta di dimissioni. So che ne avremo altre. La coalizione in quest'Aula ha il problema che le mancate dimissioni dei membri del Governo sono un rischio molto serio per noi, forse quasi più del dibattito sull'Afghanistan. Credo però che, come eletti del popolo, come parlamentari, dobbiamo valutare attentamente il diritto alle dimissioni, specie quando un nostro collega, per il pudore dovuto ai sentimenti, per il pudore dovuto ai propri accadimenti personali, non esplicita fino in fondo, giustamente, data la necessaria riservatezza, le motivazioni e la sua esigenza. Ci saranno tempi per i giochi della politica, ci divideremo su altre dimissioni che sono, appunto, politiche.

le vicende della propria determinazione storica. Quindi, nella speranza che l'ottimo capogruppo Russo Spena non ci rifaccia un altro necrologio stile Terza Internazionale, invito tutti a votare a

Credo occorra tenere ben distinte la questione delle dimissioni del senatore Malabarba da quella relativa ai membri del Governo.

ma esiste un'altrettanta profonda diversità di opinioni tra noi e lo stesso senatore Malabarba. Questo però non può far mancare il rispetto per la scelta di una persona.

Signor Presidente, desidero ringraziare il senatore Quagliariello per avere introdotto un argomento che è "l'argomento"

dovrebbe anche riflettere giacché una delle ragioni, anzi la ragione essenziale, per la quale chiediamo all'Aula di accogliere anche le dimissioni presentate dalla senatrice Turco, è data dal fatto che - come è ben noto - i componenti del Governo non possono partecipare alle sedute di Commissione. Di conseguenza, la loro partecipazione ai lavori del Senato, la loro collaborazione e cooperazione viene e cooperazione viene fortemente depressa da questo difetto di partecipazione ai lavori delle Commissioni che sono un po' il cuore della nostra istituzione parlamentare. Non conosco l'organizzazione dei lavori dell'Assemblea nazionale francese e non ricordo nemmeno quale fosse all'epoca alla quale si è riferito il senatore Quagliariello, menzionando il dibattito che in occasione della quinta Repubblica francese si accese esattamente su questo punto. Devo dire che che l'impegno a fare in modo che la partecipazione dei senatori e dei deputati al lavoro della Camera e del Senato fosse piena e avesse piena esplicazione nei lavori delle Commissioni era un principio che avevamo annunciato come coalizione in epoca precedente ai risultati elettorale. Voglio sottolineare con molta forza che, però, tutto questo non costituisce un precedente, nel senso che credo che proprio la questione sollevata dal senatore Quagliariello dovrebbe essere una di quelle che, nell'ambito di una riflessione sul nostro sistema istituzionale e sulla sua riforma, potrebbe appassionare le forze politiche molto più di quanto non lo possa fare una assolutamente comprensibile strumentalità politica che rifiuta l'accoglimento delle dimissioni di componenti del Governo, ovviamente confidando di danneggiare in questo modo la maggioranza, essendo fatto solare, noto a tutti, che la maggioranza in questo ramo del Parlamento è una maggioranza di poche unità di voto. Signor Presidente, il Gruppo UDC ha seguito molto la vicenda della richiesta delle dimissioni dei colleghi senatori.

non credo sia stato il medico ad ordinare alla collega Turco di fare il Ministro; credo abbia avuto soltanto il compito di fare il senatore, il Ministro è venuto poi per ragioni che noi non conosciamo. Da questo punto di vista, non siamo tenuti a salvaguardare i Ministri rispetto ai senatori. Siamo tenuti a salvaguardare le ragioni personali rispetto a quelle politiche. Il collega Malabarba ha posto ripetutamente la sua come questione personale. Il Gruppo UDC ha chiesto di votare soltanto la questione Malabarba distinta dall'altra e da questo punto di vista ci atterremo. Non diamo istruzioni vincolanti di Gruppo. La libertà di coscienza è una regola generale per i senatori appartenenti al Gruppo UDC. Do per scontato che questa libertà di coscienza la useranno, avendo preso presente che il Gruppo ha ritenuto di votare la questione Malabarba separatamente da tutte le altre. *(Applausi

I senatori favorevoli ad accogliere le dimissioni premeranno il tasto verde al centro della postazione di voto; i senatori contrari premeranno il tasto rosso a destra; i senatori che intendono astenersi premeranno il tasto bianco a sinistra. si tratta di uno scrutinio segreto, qualunque sia la scelta di voto effettuata, la luce che si accenderà sarà di colore neutro. Dichiaro aperta la votazione.

(Applausi).* Personalmente mi dispiace, perché ho apprezzato il collega Malabarba per tanto tempo e vanno a lui, anche a nome della Presidenza, i ringraziamenti per il lavoro svolto.

deve lasciare l'Aula. Lo salutiamo, gli facciamo molti auguri, ma deve lasciare l'Aula; non c'è, inoltre, il sostituto del senatore Malabarba. pertanto riunire a Giunta, stabilire chi è il primo nei non eletti, metterlo in condizione di partecipare alla seduta; quindi, non possiamo procedere alle dimissioni

Senatore Matteoli, è proprio nel senso da lei indicato che avevo chiesto di poter incontrare i Capigruppo. Personalmente, do una interpretazione identica a quella che dà lei, perché, comunque, deve essere garantito il *plenum* del Senato prima di poter procedere a qualunque altro atto.

Presidente, intervengo brevissimamente e solo per completezza dell'informazione. Siccome il sistema elettorale è appena cambiato in questa legislatura e l'ultimo sistema era quello maggioritario, finora era impossibile attuare questa procedura perché ci volevano mesi. la questione *pro futuro,* perché ci sono comunque sei senatori del Trentino-Alto Adige e quello della Valle d'Aosta eletti ancora con il sistema maggioritario;

Presidente, mi scuso, ma credo che nelle decisioni che stiamo prendendo ci sia qualcosa che decisamente non funziona. Dobbiamo chiederci se è fondata la decisione che stiamo assumendo ora e cioè che il Senato non possa deliberare su un punto all'ordine del giorno perché manca il suo *plenum*. Tale tesi è, a mio giudizio, assai discutibile e vi sono precedenti in cui il Senato ha proceduto in altra direzione. Sono sinceramente stupito

Senatore Morando, è evidente che la seduta pomeridiana mai potrebbe avere inizio o l'Aula deliberare se non interviene un pronunciamento della Giunta

mi sembra che vi sia un po' di confusione, perché bisogna intenderci su cosa significhi *plenum*.

Qualcuno la pensa in un modo, qualcuno in un altro, ma stiamo attenti a non costituire, con la discussione di oggi, un pericoloso, direi devastante precedente, su una questione che interessa la scienza costituzionalista

pienamente legittimata, altrimenti dovremmo buttare a mare i cinque anni della legislatura precedente, in cui la Camera dei deputati ha regolarmente deliberato con undici componenti in meno. E stiamo attenti, colleghi, perché basterebbe una Giunta delle elezioni a bloccare l'operatività del Parlamento di un Paese democratico. È un rischio gravissimo. ci misureremo sulla questione, anche con i tatticismi che ciascuno di noi cercherà di mettere in campo per portare acqua al proprio mulino, ma stiamo attenti a non mettere in discussione questo principio.

credo che se in quel momento fu espresso un voto dall'Assemblea della Camera dei deputati, la Camera fosse titolata a votare perché diversamente non avrebbe potuto farlo. In maniera molto più pratica, devo rilevare che se qualcuno avesse detto che l'Aula non era più titolata a votare finché non fosse stato reintegrato il *plenum*, anziché impiegare cinque anni si sarebbero impiegati cinque minuti per risolvere un problema che è rimasto senza